G1.32, G1.36, G1.203 (testo 2), G1.41 (testo 2), G1.1 (testo 2), G1.2 (testo 2), G1.3 (testo 2), G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2), G1.102, G1.103 (testo 2), G1.104 (testo 2), G1.105, G1.106, G2.1,

G1.202, G1.32, G1.36, G1.203 G1.203 (testo 2), G1.41 (testo 2), G1.1 (testo 2), G1.2 (testo 2), G1.3 (testo 2),

G2.1, G4.2 (testo 2) e G4.101 (testo 2) accolti dal Governo chiari, signor Presidente.

Signor Presidente, ci apprestiamo a votarlo; per cui, prima di votarlo, chiedo di leggerlo, perché non mi mette nelle condizioni di poterlo votare.

credo che sia il G1.1.01. Chiedo una verifica, cortesemente, prima di darlo per approvato.

che non ci consentono di lavorare. Basta adesso!

Vincenzo Cerami era davvero un uomo straordinario. Ha avuto una vita ricchissima. È stato molte cose nella sua vita. Non è vero che abbia soltanto fatto lo scrittore e lo sceneggiatore: ha anche lavorato in America in campi del tutto diversi da quelli letterari. Era un cittadino del mondo, un intellettuale di altissimo valore, uno scrittore - voglio ricordarlo - che ha iniziato il suo percorso con Pier Paolo Pasolini, che è stato uno dei suoi professori, quello che lo ha gli ha dato il coraggio anche di iniziare quella vita di scrittore che è stata sempre improntata, come diceva lo stesso Cerami,

di questo fatto dobbiamo ringraziare tantissimo Vincenzo Cerami. Ma Vincenzo Cerami aveva anche un lato di passione civile e di impegno politico. Io l'ho conosciuto personalmente in quella occasione: lui è stato per un po' di tempo responsabile cultura, come si suol dire, del nostro partito, il Partito Democratico. Ebbene, io non ho mai conosciuto un responsabile cultura così poco responsabile cultura, perché ci metteva tutta la vita.

mi offri?». Era un uomo che amava tantissimo la vita, era un gaudente: gli piaceva mangiare bene e bere, gli piaceva stare in compagnia e comunicare. Da questo credo abbia tratto anche la grande, straordinaria forza

tantissime cose. Dico solo che Vincenzo Cerami è stato l'intellettuale che tutti noi vorremmo poter frequentare e conoscere, ed è vero quello che dice Roberto Benigni: è un dono averlo incontrato. Lo dico in modo sincero e commosso perché, anche dal punto di vista umano, raramente una persona di così alta cultura è stata in grado di comunicare umiltà e intelligenza, con quello sguardo chiaro così ironico e così profondo che diceva tantissimo. Mi resta un rimpianto. Lui ha sempre detto: con te bisognerebbe andare a fare un tango sul Tevere. È un'immagine che trovo molto bella, perché ritrae un uomo votato alla vita e questo - ripeto - è un piccolo rimpianto che mi rimane. Ma il grande riconoscimento che voglio fare a Vincenzo Cerami sta nella sua capacità di aver associato nei suoi scritti e nelle sue sceneggiature la piccola storia degli individui con la grande storia dell'umanità, riassunto in quella semplice frase che c'è alla fine di «La vita è bella», quando il bambino abbraccia la madre e dice: «Mamma, abbiamo vinto». In quella frase c'è tutto: c'è la felicità immensa di un'umanità liberata con dietro il dolore straziante delle vittime che per la libertà hanno combattuto. Ciao Vincenzo, non ti dimenticheremo.

per la sua grande capacità di essere un affabulatore, sempre però sobrio, sempre però in grado di mettere in evidenza l'umanità profonda: quella che, appunto, si legge nell'interlocuzione con l'altro. Le sue narrazioni, sempre improntate a dare del paesaggio una grande e straordinaria vitalità, erano prima di tutto

la sua capacità di rappresentare la nostalgia come qualcosa fortemente insito nell'uomo e che connota l'umanità intera, con un ulteriore particolare che è giusto che io, uomo del Sud, metta in evidenza: il suo essere meridionale, ma non solo dal punto di vista geografico, perché la sua meridionalità rappresentava tutti i meridioni e tutti i sud del mondo.

La Presidenza naturalmente si associa al ricordo di una delle personalità più importanti del mondo della cultura e della creatività italiana.

a coinvolgere la Commissione nell'ambito delle procedure volte all'emissione di provvedimenti soppressivi di eventuali sedi o presidi delle forze dell'ordine. Trattandosi di un impegno semplicemente a rendere edotta la Commissione affinché possa dare un contributo fattivo, chiediamo che l'Aula si esprima favorevolmente, perché ci sembra un passaggio utile per avere una visione d'insieme rispetto alla lotta alla criminalità organizzata.

**Il Senato non approva**.

ordine del giorno non sfugge neanche al Governo e in questo senso abbiamo ricevuto prima rassicurazioni in tale direzione. Credo che si tratti di una riformulazione che comunque impegna il Governo in maniera forte

ci possiamo porre, considerata la delicatezza della questione e anche l'interesse ad avere presidi di questo tipo in un'area sensibile per i progetti che si stanno avviando in quella zona.

Signor Presidente, sperando che il mio intervento non turbi o non commuova anche oggi il cittadino senatore Crimi, vorrei fornire una sola delucidazione al senatore Giarrusso in ordine all'emendamento

questa disposizione con quella di cui al successivo comma 4, nel quale il regime del segreto istruttorio od investigativo - senz'altro importante, ma non

che, ove si intenda raggiungere la non opponibilità di qualsivoglia tipo di segreto alla Commissione, debba necessariamente essere ricompreso nell'emendamento da lui presentato anche il segreto di cui

di sei mesi, addirittura non prorogabile. Pertanto, non è un'opposizione netta e inevitabile, ma è un'opposizione temporanea che può anche essere

non voglio definire - di votare per persone assenti. È una cosa fondamentale anche per lei, signor Presidente, e per tutti i colleghi: è offensivo nei confronti di questa Aula votare per una persona assente. assente. Lo chiediamo in modo sereno, però poniamo fine a questa pratica ignobile! Grazie

alcuna modificazione rispetto al testo che è stato esitato dalla Camera dei deputati, perché questo consente un immediato insediamento della Commissione parlamentare antimafia:

l'opinione pubblica e i cittadini tutti si attendono risposte molto serie e concrete dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata. È una criminalità organizzata sempre più sofisticata, che sempre più ci appare vicina al mondo economico e finanziario, una criminalità organizzata prepotente e che crea le condizioni...*(Brusìo)*.

dell'allontanamento rispetto al comune sentire: oggi sempre più larghi strati della popolazione avvertono il fenomeno malavitoso della criminalità organizzata della cittadinanza stessa e come nemico delle prospettiva di crescita. Oggi il binomio criminalità organizzata‑sottosviluppo è entrato nelle corde e nel sentire della gente, nei ragionamenti quotidiani, soprattutto delle nuove generazioni e di larghissimi strati della società. Oggi sappiamo che la criminalità organizzata non uccide soltanto persone, ma uccide speranze: di prospettiva, di crescita, di futuro. Ci auguriamo che anche le note polemiche che sono apparse nel dibattito di queste due giornate possano non albergare nella Commissione parlamentare antimafia, perché deve essere la Commissione dove tutti cercano di dare il proprio contributo, al di là dello schieramento politico di appartenenza, al di là del lato dell'emiciclo dove ci si siede: una contrapposizione in quel caso sarebbe davvero assurda. Eppure è stato sgradevole dover ascoltare in quest'Aula che qualcuno ancora si attarda a voler discriminare e distinguere tra chi favorisce e chi non favorisce l'attività o le azioni della malavita organizzata. Non può esistere: tra le precondizioni della politica e del far politica il considerare questi fenomeni come davvero nemici di una società civile. Ci rallegriamo veramente anche della maturità del dibattito, che ha portato al ritiro di alcuni emendamenti che avrebbero potuto

e colleghi - che taluni emendamenti fossero presentati per il piacere o nello spirito di aprire anche ambiti di indagine sugli stessi organi inquirenti, sulle stesse persone che hanno dovuto svolgere - e coraggiosamente hanno svolto - indagini in procure importantissime e molto sensibili. Io appartengo ad una terra che ha pagato un altissimo prezzo di sangue nella lotta alla mafia. La mafia

la serenità nel dibattito, il non inserire elementi di turbativa in una lotta che non può avere né esitazioni né doppi giochi mentali, è un onore che viene tributato anche a coloro che hanno vissuto con onestà intellettuale, con grande passione e grande amore. Sono questi uomini, e concludo, signor Presidente, che devono essere devono essere di esempio, non solo per la classe politica ma per ciascun cittadino, e devono essere sempre ricordati: ricordati non per la storia che hanno costruito, ma per la storia che ancora dobbiamo costruire nella direzione della liberazione dalle associazioni mafiose di qualunque tipo. Oggi più che mai, da questa Camera alta del Parlamento italiano, deve venire un monito chiaro; lo stiamo già esprimendo con la celerità del varo della Commissione; dobbiamo confermarlo

Questo deve essere il grande messaggio morale che viene oggi dal Senato della Repubblica; questo mi auguro possa essere, con il voto unanime del Senato, il viatico della nuova Commissione antimafia, alla quale auguriamo un proficuo lavoro.

una preoccupazione che il dibattito di ieri in qualche misura ha evidenziato. La mafia non può essere questione che viene utilizzata dall'una o dall'altra parte per una lotta politica:

è necessario avere uno strumento efficace, rapido e attento, in particolare, al fenomeno, non interessato a sviluppare campagne di lotta politica, che francamente in questo momento non hanno bisogno di essere incrementate. Credo che la Commissione antimafia debba, in particolare, sviluppare l'analisi dei nuovi fenomeni, avere capacità di approfondimento effettive, sviluppare correzioni e modifiche del nostro sistema ordinamentale, che consentano una maggiore efficacia nella lotta, in particolare per quanto riguarda la tempestività di adeguamento delle nostre norme all'indiscussa capacità di evolversi della mafia verso nuovi modelli e nuove azioni. Gli ambiti di lavoro della Commissione saranno sicuramente quelli tradizionali, ma non bisogna tralasciare l'approfondimento verso nuove modalità e nuovi aspetti. In questo senso, anche le sollecitazioni che venivano dal Gruppo Movimento 5 Stelle in merito ad una visione internazionale, che tenga conto anche degli aspetti geopolitici dell'azione della mafia, rappresentano sicuramente un elemento di grande importanza. All'interno di ciò, inserisco la necessità di un approfondimento delle questioni relative all'immigrazione illegale, che sicuramente hanno contatti molto stretti La Commissione antimafia, però - devo dirlo con estrema franchezza e anche con qualche preoccupazione - deve essere presidio di garantismo; deve avere la capacità di sviluppare dibattiti ed approfondimenti che non generalizzino, ma che siano in grado di distinguere ed assegnare competenze e responsabilità, che spesso, nel passato, non sono state individuate con efficacia e puntualità. È opportuno prendere in esame anche le nuove modalità con cui la mafia fa i suoi affari, non sempre riconducibili in prima istanza al codice penale. Ormai c'è una mafia che agisce all'interno del mercato legale, coperta in particolare da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali. È quindi verso questa azione che bisogna aumentare la nostra capacità di analisi, di approfondimento e di osservazione libera dai pregiudizi, perché non si può fare la lotta alla mafia con il pregiudizio: bisogna affrontare questo argomento e questa situazione con determinazione, con ampia visione e senza verità

abbiamo molto insistito affinché il testo rimanesse quello votato alla Camera, così da avere tempi quanto più rapidi possibile. Del resto, com'è stato detto più volte nel corso di questa discussone, le attività criminali connesse alle mafie si intrecciano sempre più con una pervasiva penetrazione nella vita economica del Paese, con una grande capacità di intessere rapporti con la criminalità internazionale, utilizzando canali finanziari per l'attività di riciclaggio delle risorse, frutto spesso di attività illecite. Quindi, non solo rimangono ferme dal nostro punto di vista le capacità classiche - per così dire - di inquinamento e di corruzione della vita pubblica, che hanno per l'appunto storicamente connotato il fenomeno mafioso,

Al contrario, come dimostrano le inchieste giudiziarie, la loro capacità pervasiva di insediarsi in tutto il territorio nazionale, finanche europeo, riuscendo a radicarsi profondamente nel tessuto economico locale - producendo quindi effetti nefasti sulla vita economica, sulla legalità della sfera politica e amministrativa e sull'ordine pubblico

che permangono anche nella politica nazionale e nella pubblica amministrazione, essendo questo il vero brodo di coltura entro cui il fenomeno mafioso si alimenta e prospera, provocando, purtroppo, danni ingentissimi alla vita democratica del Paese e anche alle libertà fondamentali dei cittadini. In questo senso guardiamo con favore alla presenza, all'interno del

Proprio per questo consideriamo - lo dico naturalmente anche ai relatori - assolutamente decisivo aggiornare il nostro punto di vista. Vorremmo soffermare la nostra attenzione su un punto di fondo. Stiamo parlando, a nostro avviso, di una nuova forma di capitalismo, efficacissimo e spregiudicato. Ormai il centro di interesse del fenomeno mafioso non è semplicemente fare soldi, come in passato, ma è anche e soprattutto come investire le risorse accumulate. Parliamo, per difetto, di una stima di 30 miliardi di euro all'anno che vengono movimentati, con un'immissione nell'economia legale di un capitale in nero che fa saltare ovviamente ogni regola del mercato, permettendo, ad esempio, alle imprese mafiose di concorrere con il massimo ribasso in tutte le gare d'appalto. Naturalmente questo capitale permette anche un nuovo tipo di investimento, forse ancora più redditizio del mercato della droga; questo nuovo investimento coincide con il grande tema dello smaltimento dei rifiuti. Personalmente - i colleghi lo sanno - vengo da una Regione, la Campania, la cui cosiddetta emergenza rifiuti nel corso di questi anni non è stata semplicemente dovuta all'incuria e all'incapacità di scegliere una strada efficace da parte della classe politica locale, che pure c'è stata e che, com'è noto, è stata giustamente punita dal voto degli elettori. Ma c'è anche qualcosa in più: c'è anche il dato, che non possiamo in quest'Aula sottovalutare neanche per un attimo, del continuo e decennale sversamento illegale di rifiuti tossici industriali, gestito direttamente dalle mafie,

come ho accennato, il policentrismo mafioso ci porta a parlare di un'unica capitale, addirittura dell'intero continente, e di un'attitudine anche delle nostre grandi metropoli del Nord di non opporsi e invece di favorire purtroppo l'infiltrazione mafiosa. Ora, noi speriamo che la Commissione possa occuparsi di tale aspetto dopo che però per anni è stato sottovalutato: l'ingerenza mafiosa Grazie sulle nuove modalità con cui si è determinato il rapporto mafia‑politica: il rapporto di reciproca convenienza e anche di reciproco inabissamento. Si pensi soltanto al numero crescente di casi di candidati alle elezioni amministrative

il fatto che pochi giorni fa la Camera ‑ naturalmente speriamo lo farà anche il Senato con la stessa forza ‑ abbia modificato l'articolo 416‑*ter*

del fenomeno mafioso. Il punto di riflessione che però pongo a voi e pongo all'Aula - ed è appunto la domanda che secondo me dobbiamo farci - è se oggi non sia semplicemente una prova di civiltà, ma anche di rapporto di forza modificato mettere in discussione quell'ordinamento. Ritengo che oggi la società civile sia più forte e meno

in cui ricorre il 25° anniversario della sua morte, Peppino Impastato, ammazzato nel 1978, proprio nello stesso giorno in cui le Brigate rosse ammazzavano Aldo Moro, e ancora oggi per noi, donne e uomini della sinistra democratica, imprescindibile punto di riferimento. Mi piace pensare a lui oggi, a lui ma anche - mi vorrei soffermare pochi secondi ad altri uomini di diverse culture politiche, Piersanti Mattarella, per esempio, Pio La Torre o Paolo Borsellino (il cui anniversario della morte, peraltro, ricorre proprio domani), persone che non avevano semplicemente ruoli diversi (anche quello), ma che avevano anche e soprattutto culture politiche differenti e che però, ciò nonostante, erano unite dalla stessa condanna e dalla stessa lotta. Vorrei che oggi da parte nostra, di quest'Aula,

della Commissione antimafia, istituzione che è una costante nel nostro panorama politico‑istituzionale, la cui presenza e il cui rinnovamento, dati i compiti molto delicati e di assoluta rilevanza che è chiamata a svolgere, si giustificano alla luce della permanente minaccia che la criminalità organizzata

poiché ad oltre 150 anni dalla sua nascita non solo lo Stato unitario italiano non è riuscito a sradicare il fenomeno, ma sta scontando il suo persistente rafforzamento e allargamento, che adesso interessano anche i nostri *partner* europei. Non c'è sovranità senza controllo del territorio e monopolio della forza legale; non c'è competitività se le imprese non possono beneficiare di un ambiente sicuro. E proprio per questo motivo la lotta alla criminalità organizzata organizzata di per sé è una misura di sviluppo per il nostro Paese, e questo va sottolineato. Non esiste democrazia là dove il voto è condizionabile e lo Stato per sopravvivere deve alimentarsi anche con il denaro tratto dalla malavita o dalle organizzazioni criminali. Quindi, il quadro di esame è davvero complesso. Risponde a realismo anche l'adattamento dell'oggetto dell'inchiesta parlamentare, che si è allargato progressivamente fino a coprire anche territori differenti rispetto a quelli di origine di mafia, camorra e 'ndrangheta - come ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, così

Questo allargamento dell'oggetto cerca di tenere in considerazione e includere anche il fenomeno delle organizzazioni malavitose straniere, purtroppo presenti ormai in maniera radicata nel tessuto del nostro Paese, responsabili di reati odiosi, come il narcotraffico o addirittura la tratta di esseri umani. Nell'esprimere quindi il mio sì, e il sì del Gruppo parlamentare di cui faccio parte, al disegno di legge in esame, desidero sottolineare alcuni aspetti sui quali auspichiamo che la Commissione in via di ricostituzione possa far luce nei prossimi mesi ed anni. La trasformazione e la finanziarizzazione del crimine organizzato ci impongono in primo luogo di prestare grande attenzione all'individuazione dei patrimoni illegittimi e, parallelamente, anche al modo in cui vengono utilizzati i beni confiscati alle persone oggetto di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Ne va garantita la destinazione sociale, comunque la si voglia declinare, a favore della collettività, anche sotto forma di maggiori risorse, ad esempio da utilizzare per le forze della Polizia, che sappiamo essere, le forze dell'ordine in generale, sempre sotto organico e carenti di risorse. Questo - lo voglio sottolineare - è stato fatto all'epoca in cui alla testa del Viminale c'era il ministro dell'interno Roberto Maroni, che per primo ha capito l'importanza di aggredire le associazioni mafiose e criminali nel loro patrimonio provvedendo alla confisca dei loro beni. Grazie a lui sono stati raggiunti risultati addirittura insperati sul fronte della confisca dei beni, con l'istituzione - lo ricordo - dell'agenzia nazionale a ciò preposta, che hanno consentito di colpire nel vivo del loro sistema di sostentamento le organizzazioni criminali. Ministro ha poi provveduto - mi ricollego a quanto detto prima dal senatore De Cristofaro - anche allo scioglimento di molti Comuni e consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Dovremo quindi verificare anche l'avanzamento per quanto riguarda la lotta al riciclaggio e al gioco d'azzardo che spesso l'accompagna. Saremo chiamati anche a valutare l'applicazione delle norme adottate per assicurare correttezza nelle procedure concernenti gli appalti. Questo riguarda, purtroppo, il territorio di moltissime Regioni. Un ulteriore terreno sensibile, infine, è quello che concerne i rapporti tra criminalità organizzata e politica. Anche noi vediamo con molto favore la previsione di una fattispecie criminosa apposita

delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Quindi, non si tratta soltanto di accertare fatti e collocarli in prospettiva, ma di discutere anche di innovazioni legislative in grado di ostacolare lo sviluppo di queste connessioni, fermo restando che, purtroppo, in questo campo non ci sono soluzioni facili, come prova la circostanza che diversi Paesi fronteggiano con misure diverse dettate anche dalle urgenze del tempo lo stesso problema. Nel mondo esistono anche situazioni estreme che per noi devono essere un monito. Cito il caso del Messico, Paese che di fatto è virtualmente sprofondato in una guerra civile combattuta ad armi impari dal Governo contro i grandi sodalizi criminali legati al mondo della droga. Noi non ci troviamo in questa situazione, ma per noi la vigilanza è essenziale e, per quanti progressi si facciano, dobbiamo sempre cercare di proporre dal punto di vista normativo e legislativo strumenti ulteriori. Questi sono quindi gli impegni di domani, ai quali si potrà dar corso solo approvando la ricostituzione della Commissione antimafia. Per questi motivi il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà convintamente a favore del provvedimento.*(Applausi Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli tessere, fa specie dover constatare che abbiamo dedicato due ore e mezza del nostro dibattito di ieri per ragionare su congiunzioni e sostantivi un argomento importante come quello dell'insediamento della Commissione antimafia, in sede di dichiarazione di voto, dover parlare con un'Aula semideserta. Mi fa piacere parlare oggi dell'insediamento della Commissione antimafia, perché vorrei prima di tutto rendere onore a due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il generale Mori e il colonnello Obinu, che sono stati posti sotto processo per aver servito questo Paese e che finalmente ritrovano l'onore che hanno meritato. Finalmente. Finalmente votiamo il disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Da subito dirò che il voto di Scelta Civica sarà a favore dell'istituzione della Commissione, così come proposta dal relatore Gotor, che ringrazio per l'accurato lavoro ricognitivo della sua relazione, e ritorno su quel finalmente iniziale. Dico finalmente perché questa Commissione va a sanare un bisogno, un bisogno che affonda le sue radici in un passato che, per incuria, negligenza, indolenza, interessi, apatia, indifferenza - metteteci pure il sostantivo che più vi aggrada - non riusciamo a scrollarci di dosso. un passato - evitiamo di nascondercelo - che ha pesato e pesa sulla nostra immagine internazionale; ha pesato e pesa sui nostri rapporti istituzionali; ha pesato e pesa sui nostri rapporti economici e finanziari e, infine, ha pesato e pesa sui nostri rapporti sociali. È un passato, insomma, che ha contribuito a dilatare il solco tra Paese legale e Paese reale, del quale il presente è amara testimonianza. Ben venga allora questa Commissione, a patto però che i Gruppi parlamentari ne abbiano grande riguardo e la utilizzino con la serietà, la scrupolosità, l'austerità, la gravità e la responsabilità che la delicatezza delle sue funzioni impongono. Dico questo continuando a ritenere, in una ostinata e cocciuta visione liberale, che il Parlamento sia e debba essere innanzitutto un presidio morale. La storia e la cronaca ci dicono che non sempre, però, è stato così. Ma a questo deve tendere il nostro sforzo, ad essere e a dare l'esempio, in un momento difficile, soprattutto adesso,

che hanno animato la cultura degli ultimi anni e - perché no - le istituzioni del nostro Paese? La sfida, allora, è soprattutto in questa Commissione. Da qualsiasi angolo la si voglia guardare, questa Commissione può influire sulla condizione del nostro Paese. Vogliamo guardarla sotto il profilo economico? 200 miliardi di fatturato dell'impresa illegale sono una cifra impressionante, se solo si pensasse per un attimo, in epoca di *spending review*, al valore degli interessi che il nostro Stato paga sul debito pubblico. Togliere ossigeno alle mafie e drenare danari alle attività illecite quanto aiuterebbe il Governo del Paese in termini di aiuti alle imprese, di posti e di sicurezza del lavoro, di concorrenza leale - penso soprattutto agli appalti pubblici - o di benessere sociale? Oppure vogliamo guardarla sotto il profilo della giustizia e del rapporto tra le istituzioni? Quale strumento migliore, allora, per creare quel clima di pacificazione tra magistratura e politica, tanto caro agli esegeti delle larghe intese? O ancora: vogliamo guardarla in termini di funzione pubblica, di credito, di alterazione dei principi di libera concorrenza, di amministrazioni locali, di forze di polizia, di relazioni internazionali? Insomma, da qualsiasi parte la si voglia guardare, questa Commissione, se correttamente istituita con uomini e mezzi, serve allo Stato inteso come istituzioni e serve al Paese inteso come cittadini. Non mi perderò, quindi, in sterili dissertazioni formali sul numero dei componenti della Commissione o sulla organizzazione degli uffici. L'articolato del disegno di legge, così normato ed emendato, è un valido strumento che il Parlamento mette nelle mani dei Gruppi parlamentari. Sta a noi ora, alla nostra sensibilità e alle nostre responsabilità, mandarci donne e uomini che, sfuggendo alle effimere mode di un'antimafia di maniera, legata all'infausta dicotomia della giustizia giusta, rendono finalmente giustizia. Ecco: che queste donne e questi uomini facciano ritrovare, attraverso la ricerca della verità, la fiducia dei cittadini e il prestigio delle istituzioni. Infine, signor Presidente, formulo un auspicio personale: che il lavoro di questa Commissione renda inattuale il pensiero di un grande e fine pesatore meridionale come Corrado Alvaro, secondo il quale la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle all'istituzione della Commissione antimafia,

nostro Paese: il fiume di denaro - la Banca d'Italia parla di 150 miliardi di euro riciclati ogni anno dalle mafie delle varie Regioni, anche straniere - è un pericolo per il nostro Paese, per l'economia, per la nostra democrazia. Non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e non pensare che con 150 miliardi di euro all'anno si possa comprare non soltanto qualche bar o qualche attività economica, ma addirittura pezzi interi della politica e dei settori della comunicazione. Accade, colleghi, accade anche in Europa; non si comprende perché questo rischio non possa verificarsi o non si sia già verificato nel nostro Paese. Abbiamo il dovere di indagare, perché il Movimento 5 Stelle pensa che per riciclare 150 miliardi di euro all'anno non siano sufficienti qualche bar e qualche pizzeria e nemmeno una filiale di una banca ci vogliono intere banche, interi consigli d'amministrazione, che non possono far finta di non sapere. Sono gli stessi consigli d'amministrazione che in questi anni abbiamo scoperto essere marci, fradici, invasi dalla corruzione, dannosi per la nostra economia,

c'è anche il riciclaggio del denaro sporco. Noi dobbiamo indagare, perché il nostro Paese non può correre questo rischio, signor Presidente. Annunciamo il nostro voto convinto anche chiedendo scusa. Dobbiamo chiedere scusa a Paolo Borsellino, a Emanuela Loi, a Vincenzo Li Muli, a Walter Cosina, a Claudio Traina. Noi dobbiamo chieder loro scusa, perché questo Stato non li ha difesi quando si sapeva che stavano per morire. Dobbiamo chiedere scusa perché, a distanza di tanti anni, non abbiamo ancora la verità su questi fatti. Noi del Movimento 5 Stelle siamo qui, mandati dai cittadini, per scoprire la verità anche su questi fatti, signor Presidente. Noi chiediamo scusa a questi uomini che hanno sacrificato la propria vita per questo Stato, perché non era questo lo Stato che loro immaginavano; non era lo Stato che consegnava una donna e una bambina a una dittatura quello per cui loro sono morti.

Signor Presidente, la domanda che dobbiamo porci è se ancora oggi ha senso una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Per noi la risposta è sì. Dal dibattito che ieri ci ha occupato, ho notato che lo spirito che questa Assemblea ha espresso è quello giusto. Da diverse esigenze culturali e politiche è emerso in maniera univoca che questa Commissione deve, anche in questa legislatura, essere costituita. Il testo è sostanzialmente quello della scorsa legislatura e non ci sembra che presenti ostacoli alla sua approvazione. Sento di ringraziare per il lavoro svolto la presidente Finocchiaro Grazie, interamente, ma anche per il suo lucido intervento di ieri, che ha consentito di evitare la navetta che nulla o poco avrebbe aggiunto al testo, già chiaro circa i compiti che devono essere alla base del lavoro della costituenda Commissione. La lotta alle mafie è compito precipuo delle forze dell'ordine e della magistratura, alle quali va il nostro più sentito ringraziamento per quello che quotidianamente svolgono, a volte con il costo della vita di chi ne fa parte e dei suoi congiunti, e anche con il costo della propria dignità, come è accaduto al generale Mori e al colonnello Obinu, ai quali vanno il nostro pensiero e la nostra solidarietà. Il compito della costituenda Commissione dovrà essere, quindi, quello di tenere sempre viva l'interlocuzione con la magistratura e con i rappresentanti delle forze dell'ordine e fare tesoro di tutti i suggerimenti, oltre che di capire i tanti *vulnera* che la legislazione vigente ancora contiene. La Commissione antimafia deve essere un interlocutore costante e un baluardo delle istituzioni affinché tenga sempre una luce accesa sulle attività criminali che distruggono il tessuto sociale del nostro Paese e la crescita civile, oltre ad inquinare la nostra società. La Commissione deve sforzarsi di guardare anche oltre le nostre frontiere, perché ormai il fenomeno criminogeno e degenerativo è globale. Oggi variamo la decima Commissione, ma già da domani dobbiamo pensare a come questa possa meglio svolgere il suo alto compito. Il voto compatto di tutta l'Assemblea sarà un grande stimolo per tutti.

Ci stiamo solo assumendo delle responsabilità; stiamo parlando della nascita di uno strumento, una Commissione, che ha compiti ben precisi, che non esautora il Parlamento ma, semmai, lo responsabilizza. Non esautora il Parlamento perché non c'è tutto quello che ci potrebbe essere. La collega,

Ci sono tante altre cose che potremmo approfondire e altre che potrebbero restare fuori dalla competenza della Commissione. Ci tengo a dire questo, perché altrimenti sarebbe troppo semplice votare una Commissione - ribadisco, uno strumento - e pensare che il Parlamento non ha più responsabilità. Qualcuno nel suo intervento ‑ mi pare fosse il senatore Lumia ‑ ha parlato dell'antimafia del giorno dopo. Certo, non è facile allontanare questa immagine e impressione. Devo dire che le Commissioni che si sono succedute altro non hanno fatto hanno fatto che adeguarsi ad una realtà che è stata in evoluzione negativa, ma anche ad una realtà che è cambiata. Certo, nel 1962, quando è nata la prima Commissione antimafia, si parlava soprattutto di Cosa nostra, non si parlava delle altre mafie; figuriamoci se si parlava delle mafie internazionali e delle mafie globalizzate, in un momento in cui Cosa nostra aveva la scena assoluta. Le cose sono evolute: ci sono oggi, anche nei confini nazionali, altre mafie, a partire dalla 'ndrangheta, che hanno guadagnato la scena e sono diventate potenti sotto il profilo dell'offensività, sotto il profilo strategico, ma anche sotto il profilo economico. Quindi c'è una mafia in evoluzione, più forte e - se vogliamo - anche più aggressiva del passato. Su questo la politica si deve interrogare, perché ha delle responsabilità.

si è osservato che la promessa di voti in cambio di denaro è un'ipotesi di reato la cui prova è quasi impossibile. Sarebbe necessaria una riformulazione della norma che, pur non lasciando alla magistratura eccessivi margini di discrezionalità interpretativa e applicativa, sanzionasse in modo efficace e non soltanto declamatorio il voto di scambio politico-mafioso». Stiamo parlando a vent'anni di distanza da questa osservazione, e l'ho richiamata perché le cose che scriviamo devono avere un senso. Esattamente vent'anni dopo la Camera dei deputati ha approvato una modifica

riconnetto grandissima importanza: nell'articolato che istituisce la Commissione è prevista ovviamente una relazione di fine lavori, ma è prevista anche una relazione annuale

perché Borsellino rappresenta, nel panorama purtroppo numeroso delle persone vittime di una morte ingiusta, dei morti per mano mafiosa, il simbolo di quella che è stata la solitudine dei magistrati che hanno lavorato su questo fronte; la solitudine di chi opera

di attesa in cui tutti sapevamo, dopo la morte di Giovanni Falcone, che toccava a Paolo, anche noi magistrati - all'epoca io ero un giovane magistrato - sapevamo che stavano per uccidere Paolo Borsellino. Guardate che la solitudine c'è anche per tanti altri magistrati, che lavorano sul fronte e hanno bisogno di essere sostenuti mentre sono vivi e svolgono il loro lavoro, mentre vengono denigrati, mentre vengono messi alla berlina da una politica che non sempre è disposta a capire *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*. Il mio pensiero va anche a quei magistrati che hanno vissuto questa solitudine, che si sono ritirati in buon ordine o sono stati messi da parte

guardate che è facile riconoscere, se si vuole riconoscere. Quando ad una ditta del Nord viene chiesta in blocco l'assunzione di dodici operai del Sud qualcuno deve guardare. Guardate: bisogna stare attenti ai soldi ed all'origine dei soldi. Il compito del Parlamento, ad esempio, è quello di bloccare

Quando voi troveremo la strada per bloccare investimenti mafiosi, al Sud come al Nord? Quando ritroveremo la strada per riprendere la competitività del nostro Paese sulla base di appalti, di lavori di opere pubbliche svolte lecitamente, se non sapremo bloccare, se non sapremo mettere questa barriera? Allora, non guardiamoci con diffidenza. Sappiamo Sappiamo che vi sono differenze fra di noi e diverse sensibilità; sappiamo anche che tra noi possono esserci persone che non la pensano esattamente così, a destra come a sinistra, perché abbiamo avuto disavventure a destra come a sinistra (forse in alcune parti politiche di più ed in altre di meno).

la modifica dell'articolo 416-*ter*, che subito si introduca il reato di autoriciclaggio, con uno scatto di orgoglio di chi vuole ricordare le persone che si sono sacrificate. E soprattutto diamo il senso, alla società civile che ci guarda e che spesso è più avanti di noi, che qui dentro non ci sono né condannati né inquisiti - e non ce ne devono essere - ma ci sono persone che si assumono la responsabilità di capire le cose da fare e di farle fino in fondo.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 93, 656, 722 e 827.

Il patron, ovviamente, perse la presidenza del Gruppo per «mancanza di requisiti di onorabilità» ma, incredibilmente, rientrò come presidente onorario. Si sa, questa è l'Italia. Così subentrò la figlia Jonella. La storia, più o meno, è nota a tutti voi: si snoda attraverso indagini su grandi appalti, accuse di falsificazioni di voci di bilancio, una gestione criminosa di *holding*, fusioni societarie e speculazioni finanziarie. Ieri mattina li hanno arrestati tutti: padre, tre figli e amministratori delegati di FONSAI. L'accusa di reato è di falso in bilancio aggravato e false comunicazioni di mercato. Sulla scia dei fatti milanesi dell'anno scorso riguardanti la Premafin è partita l'indagine su FONSAI dalle denuncie di piccoli azionisti. Il problema principale è questo: c'è un sistema famiglia che, grazie alla complicità e al coinvolgimento di banche e politici, di finanza e mafia, alla cecità dei controllori ISVAP e CONSOB, riesce a distrarre centinaia e centinaia di milioni di euro facendo fallire le società che amministra (2 miliardi di euro di perdite, ma sempre con buonuscite milionarie per gli amministratori). Questo succede da trent'anni. Anche nell'ultimo tentativo di salvataggio voluto da Mediobanca, tramite una fusione tra grandi debitori (FONSAI e UNIPOL), ci hanno rimesso i risparmiatori, gli azionisti che nel 2011 e nel 2012 non hanno ricevuto dividendi e hanno perso il 90 per cento Ci hanno rimesso i lavoratori licenziati e quelli che rischiano il posto di lavoro e, ovviamente, i gruppi assicurativi che in passato erano considerati grandi eccellenze italiane. Ricordo al Governo che molte società intestate alla famiglia sono coinvolte nei lavori dell'Expo 2015. Pretendiamo un rigoroso controllo e la dovuta trasparenza. Chissà perché, noi non ci fidiamo. Questo sistema di collusioni deve finire. I cittadini chiedono giustizia per il danno economico e morale. Qualcuno in borsa ha commentato che è più difficile perdere soldi nelle assicurazioni che farne. Eppure, i Ligresti ci sono riusciti. Dirò di più: Alberto Nagel, il direttore di Mediobanca, interrogato dagli inquirenti ha detto che don Salvatore aveva minacciato di suicidarsi se la banca non avesse tenuto fede alle promesse da lui pretese. Sarebbe stato bello se anche in altre casi le banche avessero avuto tale attenzione per tutti i cittadini. Forse, ci sarebbero stati meno imprenditori e lavoratori

Signor Presidente, è notizia delle ultime ore la perquisizioni da parte della Guardia di finanza nella sede della fondazione VeDrò, pensatoio *bipartisan* - come adesso va di moda dire - cui fanno riferimento Enrico Letta, Angelino Alfano e altri Ministri e politici: da Orlando, De Girolamo, Lupi, l'ex ministro Idem, passando per il sindaco di Firenze Renzi, i leghisti Tosi e Giorgetti, per poi tornare nuovamente a Boccia, Mara Carfagna, Renata Polverini ed altri. La Guardia di finanza, nell'ambito di un'inchiesta sul consorzio Venezia Nuova e su quell'ecomostro che è il Mose, ha perquisito la sede romana della fondazione e anche l'abitazione a Perugia di Riccardo Capecchi, tesoriere della suddetta fondazione (anche se non risulta per nulla indagato), ma anche stretto collaboratore del Presidente del Consiglio, appunto, Enrico Letta. Sotto indagine sono le sponsorizzazioni per decine di migliaia di euro del consorzio Venezia Nuova che ha sponsorizzato anche, ma non solo, la fondazione di Enrico Letta e Alfano. Il Movimento 5 Stelle, già in tre occasioni in Parlamento e con apposite interrogazioni, ha denunciato come occorra velocissimamente maggior chiarezza e trasparenza nel rapporto tra le fondazioni politiche e i loro *sponsor*, legittimi nella misura in cui, appunto, sono chiari e trasparenti. Lo si è denunciato alla Camera il 29 aprile per l'insediamento del Presidente del Consiglio, ha detto che la fondazione VeDrò riceve finanziamenti da aziende importantissime, in cui lo Stato ha quote azionarie rilevanti, come appunto ENI ed ENEL. Lo abbiamo nuovamente fatto al Senato, con il collega Giovanni Endrizzi, il 22 maggio, denunciando i rapporti tra le società del gioco d'azzardo, tra cui Lottomatica e Sisal, e la politica, inclusa la fondazione VeDrò. Lo abbiamo ribadito nuovamente in Senato, in data 30 maggio, con la collega Paola Nugnes, facendo luce sempre su VeDrò, la fondazione di Letta e Alfano, e i vari *sponsor* economici e politici. Di fronte alle perquisizioni delle ultime ore e alla grande influenza politica di questa fondazione e dei politici chiediamo che il Parlamento non indugi più e che chieda il più rapidamente possibile al Presidente del Consiglio quanto meno di garantire trasparenza, evidenza e solarità, perché sul finanziamento della politica e delle fondazioni i cittadini italiani penso abbiano diritto a sapere come stiano le cose. Pertanto, domani mattina si voteranno le dimissioni di un Ministro che appartiene a questa fondazione. questo nome «VeDrò», che deriva dal verbo «vedere», permetta a tutti quanti gli italiani di poter vedere nel merito se quanto oggi è oggetto di indagine sia effettivamente pulito, onesto e trasparente, oppure no.

un attacco diretto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli interni rispetto a un problema che è molto serio. Richiamando la discussione che abbiamo avuto sulla mafia, io ho ricordato che Falcone amava

questa azione del Movimento 5 Stelle che in piazza ha manifestato contro il finanziamento pubblico ai partiti, tentando anche di evitare un finanziamento per il 2013 che serve per pagare i dipendenti e le spese che i partiti hanno sostenuto in campagna elettorale. Quindi, seguendo questa teoria,

alla possibilità che le fondazioni, visto che non c'è il finanziamento pubblico, possano ricevere dei contributi. Ma da parte di chi? Se cancelliamo il finanziamento pubblico, chi può finanziare le fondazioni e i partiti? Evidentemente i privati o lo associazioni. Allora basta che una fondazione seria, di cui fanno parte personaggi autorevoli, riceva una visita della Finanza, che già si traggono le conclusioni politiche e si mette in discussione il ruolo del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno.

che sono stati commessi reati da parte di quelle imprese veneziane, perfetto: pagheranno quando sarà accertata la loro responsabilità. Ma che in Parlamento, al Senato, per una ispezione della Guardia di finanza, si arrivi già alla conclusione di mettere sotto accusa mezzo Parlamento e mezzo Governo, la considero una cosa barbara e indegna. Non faccio finta di non sentire, respingendo al mittente queste accuse.

le fondazioni finanziano i partiti, ma del finanziamento alle fondazioni - che è, quindi, la fonte

Chiediamo da tempo che sulle fondazioni si faccia chiarezza, che le fondazioni rendano pubblico da chi ricevono i fondi che poi dirottano ai partiti. *(Applausi

in un sito che si intitola «Timoretremore» si commenta e si contestualizza questa frase di Giovanni Falcone.

«Il sospetto (diceva Giovanni Falcone che il sospetto è "l'anticamera della calunnia") e la diffidenza verso tutto ciò che è al di fuori dalla nostra "normalità" (forse il nostro stile di vita è l'unico possibile solo perché non abbiamo la capacità di vedere oltre...) sono entrati in modo prepotente a far parte della nostra vita quotidiana. E in politica, dove sospetto e diffidenza sono di casa, è più facile (e comodo) ottenere consensi con l'esclusione e la paura piuttosto che con l'accoglienza, la partecipazione e la solidarietà». Questo era il contesto.